tentando di recuperare le ragioni che confermano la sua assoluta coerenza con recenti provvedimenti con recenti provvedimenti che questa Aula ha approvato e che l'altro ramo del Parlamento ha in fase di esame. Entro quindi nel merito. Parliamo della costituzione di nuovi ordini professionali e di albi inseriti nell'ambito di nuovi ordini professionali.

patrimonio di esperienze, di idee e di ideologie di ciascuno dei colleghi parlamentari, in particolare di quelli che sono intervenuti. Credo che un punto sul quale vale la pena intrattenersi, perché rappresenta probabilmente lo spartiacque del ragionamento, riguarda la necessità di ricordare che vi è una diversità fra l'attività professionale

la normativa si è innovata con riferimento a quanto di recente noi abbiamo approvato con l'ultima manovra che oggi riceverà il via libera dalla Camera dei deputati. Tuttavia, va ricordato che l'attività professionale non può rispondere solo alle logiche del mercato, né da esse può essere condizionata, tenuto conto della peculiarità della professione intellettuale, nell'ambito della quale il professionista per definizione

e la prestazione del professionista è una prestazione di mezzi e non di risultato. Va, dunque, precisata e ribadita la distinzione tra professioni intellettuali e attività d'impresa, ricordando che l'attività professionale viene svolta nel rispetto delle norme deontologiche, a tutela del soggetto nell'interesse del quale la prestazione è resa e secondo i principi della responsabilità, dell'autonomia, della indipendenza e dei profili di responsabilità diretta ed individuale dell'erogatore della prestazione stessa. Il punto è questo: vogliamo omologare le norme che sovrintendono alla disciplina delle attività delle professioni intellettuali alle logiche del mercato, oppure, pur aprendo - come peraltro è già accaduto nel passato (mi riferisco soprattutto alla legge Bersani)

esclusive di profitto sulla spinta dei processi di globalizzazione che premiano le logiche del mercato a possibile detrimento di una dimensione etica, di appropriatezza, di efficienza e di efficacia, che sono le cifre distintive che devono accompagnare l'atto professionale erogato dalla professione intellettuale?

sostanzialmente le disposizioni contenute all'articolo 3 della manovra finanziaria in fase di approvazione, nel senso che fanno propri i principi i principi richiamati dall'articolo 3 in ordine agli obblighi previsti, dove si considera che entro i 12 mesi successivi all'approvazione tutti gli ordinamenti professionali devono essere riformati al fine di eliminare ogni tipo di restrizione o vincolo che possa determinare nocumento allo sviluppo della concorrenza e del libero mercato. Vorrei ricordare che esiste una

professioni oggi riconosciute ma che svolgono la propria attività nell'ambito del comparto sanitario,

che il provvedimento affida agli statuti, approvati previa verifica da parte del Ministero vigilante,

democratico alle operazioni di voto per la rappresentanza degli ordini, i principi generali che disciplinano la tutela delle minoranze, minoranze, i principi in ordine alla modalità di accertamento dei saperi, quindi sul versante della formazione. Vengono altresì stabiliti, in uno specifico articolo, i requisiti che consentono l'iscrizione. Anche in questo caso verifichiamo l'assoluta assenza di vincoli e restrizioni per chiunque sia in possesso del titolo di laurea, conseguito in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione. Invece, avendo conseguito il titolo in uno dei Paesi

Vengono altresì stabiliti come obbligatori i principi di trasparenza delle azioni intraprese dall'ordine, i principi di leale collaborazione con lo Stato, la separazione delle funzioni di indirizzo politico dalla gestione amministrativa. Insomma, un insieme di norme che

dove - ricordo ancora una volta -è previsto espressamente che gli ordinamenti professionali vengano ammodernati, ristrutturati, rinnovati nel loro attuale assetto, ispirandosi ai principi di abolizione di vincoli e di restrizioni e svolgimento di funzioni di carattere pubblicistico orientati alla tutela della collettività. Si rilancia così la funzione dell'ordine professionale, non soltanto in termini formali ma sostanziali, per quel che realmente è: una funzione di tipo pubblicistico che tenta a fatica - e direi anche tardivamente - di scrollarsi di dosso quei residui di corporativismo che forse è il punto principale di debolezza che desta perplessità in ordine alla riconoscibilità di questi enti, che vengono percepiti soprattutto come strutture corporative, con funzione autoreferenziale, tendenti a disciplinare gli accessi nel mercato del lavoro in modo protettivo e non aperto. Questi sono i punti di debolezza che vanno rimossi. Ed io sono fortemente convinto dell'assoluta necessità che questi enti continuino ad esistere, che svolgano le loro funzioni attraverso un apparato normativo capace di rigenerarsi e di ristrutturarsi, essendo in quasi tutti i casi un sistema normativo datato. Parliamo degli ordini delle professioni sanitarie ed entriamo un po' nel merito. L'impianto normativo risale al decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato del 1946.

Sulla base di questa assoluta carenza normativa, di questa lacunosità che nel corso dei decenni si è venuta a determinare per un mancato adeguamento delle norme di disciplina di questi enti, noi non possiamo affermare e consolidare il principio per cui gli ordini sono solo un elemento di vincolo per lo sviluppo della concorrenza e del mercato. Noi dobbiamo dire che gli ordini devono esistere, ma dobbiamo farli funzionare attraverso una revisione complessiva delle disposizioni che ne disciplinano l'attività.

perché l'ordine degli infermieri e quello delle ostetriche sono sostanzialmente un cambio lessicale, perché già dal 1946, con la legge istitutiva degli ordini e delle professioni sanitarie, furono istituiti gli ordini dei medici, dei farmacisti, dei veterinari e i collegi degli infermieri e delle ostetriche con medesime prerogative, medesime modalità di funzionamento, con un regolamento di attuazione, quello del 1951, identico per tutti i cinque profili professionali, di modo che oggi noi cambiamo la parola "collegio" con l'altra "ordine". La natura giuridica resta la medesima: erano enti non economici ausiliari dello Stato, restano configurati con la medesima classificazione. Quindi, parliamo di tre ordini professionali. Né deve turbare il fatto che si istituiscano 20 e più albi professionali, perché gli albi sono degli elenchi. Tutt'al più, bisognerebbe essere soddisfatti di dare disciplina organica ad attività intellettuali dell'area medica medica che meritano di essere codificate attraverso leggi, essendo attività che si svolgono da diversi decenni in modo non regolamentato. La deregolamentazione, in generale, non rappresenta un presupposto che agevola la concorrenza e il mercato. Se la regolamentazione non è costretta e compressa dentro vincoli e restrizioni inaccettabili, è una condizione di disciplina che garantisce la comunità. E quando la prestazione riguarda atti che si riferiscono alla tutela della salute, io credo che non solo sia giustificata, ma sia opportuna e addirittura necessaria. Così come necessaria è questa legge, che evita che nel nostro Paese possano esserci professionisti della sanità di serie A e professionisti della sanità di serie B. Sono circa 500.000 gli operatori che oggi trovano dentro questa legge la riconoscibilità di una funzione ma, soprattutto, la regolamentazione della loro attività determinandosi evidentemente non solo attraverso il coordinamento dei testi di precedenti disposizioni, un quadro normativo chiaro, e determinandosi anche le condizioni perché si superi la disparità tra vecchie e nuove professioni, sia rilanciata la funzione degli organismi rappresentativi delle professioni, anche in questo tipo di attività si possa svolgere un'attività di verifica e controllo che è il migliore antidoto per combattere l'abusivismo professionale, del quale resta vittima una platea estesissima di pazienti nel nostro Paese. introduce il principio della terzietà nel procedimento disciplinare e, come dicevo poc'anzi, attraverso gli statuti viene previsto l'obbligo di rispettare quanto è stato stabilito dall'articolo 3: quindi, non c'è nessun contrasto. Anzi, io ritengo che vi sia un'assoluta coerenza con le disposizioni di legge che noi stiamo per approvare alla Camera, ma anche con quanto stabilito dall'Atto Camera n. 4274, avente ad oggetto la normativa in materia di sperimentazione clinica e di riforma, dove, all'articolo 6, è data la delega al Governo dei vecchi ordinamenti professionali per evitare che vi sia un'asimmetria un'asimmetria tra questi che oggi noi discipliniamo con norme che tendono alla modernità e, invece, i vecchi ordini professionali che sono ancora asfittici nella normativa che li disciplina. Quindi, bene ha fatto il Ministro della salute a prevedere un'apposita delega, che la Camera dei deputati in Commissione ha licenziato, e che io auspico possa arrivare in Aula

gli elementi di riscontro a quanto stabilito dall'articolo 3 della manovra finanziaria in riferimento alla liberalizzazione delle attività professionali. Penso ci siano tutte le motivazioni per una riflessione più serena, evitando, Presidente, la spinta della globalizzazione e le logiche del mercato finiscano con il prevalere rispetto ad una norma che è scritta in modo attuale e coerente e che non è assolutamente antitetica

ci sono alcuni elementi di questo disegno di legge che non soltanto non convincono ma che, testimone ne è l'ultimo intervento, cercano di interpretare altre decisioni recentemente assunte del nostro Senato che vanno in una direzione diametralmente opposta da quella poc'anzi riportata dal senatore D'Ambrosio Lettieri. Ci troviamo - credo che in via incidentale occorra segnalarlo di fronte ad un provvedimento che va a creare dei nuovi ordini e dei nuovi albi (poi magari bisognerebbe ricordare quali sono, perché se non vi è dubbio che alcune delle professioni

economici molto importanti. Le Commissioni che di queste due questioni si interessano precipuamente sono la 1a e la 5a, che sono state coinvolte per i pareri, ma che credo avrebbero dovuto essere coinvolte anche durante la preparazione Il senatore D'Ambrosio Lettieri ha detto poco fa che non vi è contraddizione con l'articolo 3 della manovra, quello che in qualche modo andava a introdurre il principio di libertà di impresa e di garanzia della concorrenza. Ecco, è difficile, anche sulla scorta degli elementi portati alla nostra discussione di ieri, comprendere come la creazione di un nuovo ordine professionale piuttosto che l'elencazione di ben 20 albi professionali possano in qualche modo andare incontro alla libertà d'impresa e alla garanzia della concorrenza. Ho anche sentito dire che occorre prima creare questi ordini per poi successivamente organizzarli e regolamentarli e quindi, magari successive norme, consentire che questi rispettino i principi, che comunque all'interno della legge già ci sono, di trasparenza, di rispetto delle cosiddette minoranze

La senatrice Poretti ieri ha esposto tutta una serie di esempi di recenti misure che, pur figlie di una proclamata necessità di apertura al mercato, di una proclamata necessità di affrontare alla radice alcuni dei problemi che negli ultimi 35-40 anni hanno fatto dell'Italia il Paese europeo con il secondo debito pubblico, accumulato grazie alle consorterie partitocratiche che pubblicizzavano le perdite e privatizzavano gli utili per gli stessi partiti politici e anche per gli amici degli amici (molto spesso imprese decotte che tutt'oggi vivono e prosperano, magari

per cortesia, sarebbe piuttosto sgradevole sospendere la seduta, ma non è possibile continuare in queste condizioni. sulla riforma della professione forense che partiva dall'assunto che occorresse limitare l'accesso alla professione e anzi, se possibile, espellere alcune decine di migliaia di professionisti perché esiste una sovrabbondanza di offerta di quel tipo di servizio; quindi, derivando da questo obiettivo centrale, ha creato tutta una serie di paletti in entrata e di criteri di criteri per cui, se non si esercita la professione forense prevalentemente, se ne viene espulsi con meccanismi che sono stati proclamati trasparenti ma che invece sono praticati «a circuito chiuso» per quanto riguarda la professione stessa. Peraltro, stessa. Peraltro, negli ultimi due mesi abbiamo adottato due manovre, in parte perché erano necessarie e in parte perché chi continua a comprare il debito pubblico italiano le ha ritenute urgenti, oltre che necessarie. In queste ore si inizia a maturare la convinzione che sia difficile sostenere il continuo acquisto del debito pubblico italiano. Tuttavia, piuttosto che riformare alla radice lo Stato sociale, piuttosto che mettere mano alla previdenza, piuttosto che cancellare le vere ruberie e i veri sprechi, si propone cosa qualunquistica tanto quanto quella del cosiddetto Parlamento pulito - da una parte di dimezzare il numero dei parlamentari e dall'altra di cancellare *ex abrupto* le Province senza neanche promuovere nel contempo le aree metropolitane o una vera e propria federalizzazione del nostro Stato; né si pensa di avviare una riforma radicale delle nostre Forze armate, che contano complessivamente oltre 180.000 persone in divisa, all'interno di un'Unione europea

riabilitative, tecnico-sanitarie, tecniche della prevenzione, alla professione sanitaria ostetrica ed equipollenti, a prescindere» - attenzione bene - «dal conseguimento del titolo di studio di istruzione secondaria superiore». Allora,

fosse esaminata maggiormente nel dettaglio, avrebbe dovuto affrontare, magari come considerazione preliminare e quindi altrettanto necessaria riforma strutturale, che ieri ha svolto il senatore Menardi, il quale ha posto l'accento sul problema dei problemi. E il problema dei problemi, ogniqualvolta si parla di una professione, è la caratteristica italiana dell'esistenza del valore legale dei titoli di studio. In pratica, con gli anni, si è ormai consolidato e - ahinoi! - cristallizato, salvo sempre fare l'eccezione di proclamarlo in campagna elettorale come qualcosa da distruggere, l'atteggiamento per inerzia culturale per cui si studia per avere un pezzo di carta piuttosto che per acquisire delle capacità specifiche, tecniche e professionali, per poi poter praticare una professione.

Anche sulla base di alcuni interventi critici o comunque di riflessione, io credo che possa essere il caso di fermarci un attimo e rinviare alle Commissioni competenti questo disegno di legge

con delle osservazioni relative al disegno di legge n. 1142, recentemente licenziato con ampia convergenza dalla Commissione igiene e sanità del Senato, per l'istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie ancora sprovviste di tale istituzione organizzativa. Questo è un provvedimento datato, su cui abbiamo avuto modo di confrontarci molto in Commissione, atteso dalle categorie rappresentative di queste nuove professioni sanitarie (nuove non tanto in quanto di recente istituzione, ma in quanto professioni sanitarie che necessitavano di un inquadramento, di un ordinamento che le trattasse oramai alla stessa stregua di altre professioni sanitarie per le quali la normativa e la regolamentazione avevano ben altre date). Questo progetto di legge, infatti, è il frutto di una meticolosa elaborazione, che contempla tutta una serie di esigenze delle varie ed eterogenee professioni sanitarie, dai tecnici di laboratorio ai fisioterapisti, ai logopedisti e agli audiometristi, i cui ambiti operativi si distinguono talora anche molto nettamente. Tra queste, la professione svolta in particolare dai tecnici di laboratorio spicca, nel contempo, per ambiti di specializzazione e consistenza numerica. I pregi del disegno di legge n. 1142 consistono, innanzitutto (sembra banale evidenziarlo, ma non lo è), nell'effettiva applicazione della legge n. 43 del 2006, voluta fortemente dal precedente Governo Berlusconi e successivamente «affossata» dal Governo Prodi, che ha fatto decadere la delega per l'attuazione dei nuovi ordini delle professioni sanitarie e, quindi, nel completamento di un lungo cammino relativo allo sviluppo su *standard* europei delle cosiddette professioni sanitarie ausiliarie o non mediche, verso una loro completa autonomia operativa e professionale, iniziato con le leggi n. 42 del 1999, n. 251 del 2000 e n. 43 del 2006, in esito al quale si potranno realizzare, finalmente, almeno quattro fondamentali obiettivi. è quello dell'applicazione di principi deontologici ed etici convalidati e resi noti a seguito di confronto con il competente Ministero, quello della salute, su proposta delle stesse professioni, con la conseguenza che ciascun operatore potrà conoscere preventivamente e in modo certo i canoni deontologici vigenti per la sua attività professionale e che ciascuno potrà essere assoggettato, in contraddittorio e nel rispetto del principio di difesa, a verifica disciplinare sugli eventuali addebiti di violazioni di tali principi, nel preminente interesse del cittadino. Il secondo punto fondamentale ritengo sia, cari colleghi, l'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo professionale, mediante la quale si permetterà al cittadino (anche via Internet, come già avviene per l'ordine dei medici e odontoiatri) di sapere che il professionista è provvisto delle competenze necessarie ed è abilitato all'esercizio della professione, e che lo stesso appartiene a una comunità autoresponsabile di colleghi, con cui si relaziona anche per la formazione continua. In questa sede, vorrei segnalare i danni fisici, psicologici ed economici dalle forme di abusivismo professionale nel campo delle professioni sanitarie non ancora regolamentate

podologi, tecnici di laboratorio biomedico e tecnici della riabilitazione che andavano a fornire prestazioni sanitarie senza alcuna competenza o titolo scientifico. Queste forme di abusivismo sono state stimate in circa 150.000 unità su un totale di 550.000 operatori censiti dal Servizio sanitario nazionale, soprattutto nell'ambito dell'attività libero professionale o di strutture private accreditate. Il terzo punto fondamentale riteniamo sia l'iscrizione all'albo come strumento che, garantendo la legittimazione di ciascun iscritto a esercitare la professione, previene la professione, previene in maniera più efficace e decisiva l'abusivismo. Inoltre, verso gli altri Paesi, in particolare dell'Unione europea, si favorisce una certezza di provenienza del professionista italiano, riguardo all'ordine del capoluogo italiano presso il quale il professionista è iscritto. Di particolare rilievo sono anche i punti del disegno di legge che tendono a tutelare l'autonomia delle singole professioni (oltre 20) nei rispettivi profili e nel loro proprio proprio campo di operatività. Infatti, attraverso le distinte commissioni di albo e la relativa organizzazione, sarà possibile salvaguardare la specificità di ciascuna categoria professionale. Nell'ambito dei

l'importantissimo ordine delle professioni sanitarie della riabilitazione e quelli dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni tecnico-sanitarie e della prevenzione. Ritengo sia fondamentale l'individuazione di questi albi, che sono di per sé una tutela

che attiene ad esempio alle tecniche di riabilitazione (che - come sappiamo - grazie soprattutto ai notevoli progressi delle scienze mediche e della ricerca

tecnici come quello della neurofisiopatologia, che possano andare ad individuare con chiarezza delle specializzazioni che per forza devono oramai distinguersi sempre più dagli altri ambiti professionali. La presenza di questi albi poi permetterà, secondo me, una migliore organizzazione territoriale (che - come sappiamo - ovviamente è gestione delle Regioni) e alla fine anche un maggiore risparmio.

di superare quella prassi, che troppo spesso avviene, di veicolare l'intervento riabilitativo con macrostrutture, macroassociazioni, macrosocietà di riabilitazione, che poi troppo spesso fanno il loro interesse, il loro guadagno, invece di liberare il singolo professionista, che allora sì diventa imprenditore di sé stesso, una volta che è riconosciuta la sua professionalità nell'albo, e andare ad essere lui stesso direttamente, così come avviene per gli specialisti medici, convenzionato con la Regione, con la ASL, con l'ente locale, in maniera che la singola Regione o ASL affidi il paziente singolarmente al nuovo professionista sanitario iscritto nel suo albo di competenza (pensiamo ai professionisti della riabilitazione), affidando a lui direttamente la presa in carico del paziente, a costi certamente più contenuti rispetto a come avviene nella quasi totalità delle Regioni a presa in carico - ripeto - di sovrastrutture di carattere troppo spesso economico, che non forniscono una prestazione diretta, ma a costi ben maggiori veicolano un'organizzazione che fa perdere solo energia e qualità Il quarto punto che volevo sottolineare è quello della formazione professionale. Noi riteniamo, anche dal dibattito avvenuto in Commissione con il presidente Tomassini e con la

dei singoli albi, che tramite questo tipo di organizzazione potranno vedere attuate quelle forme di sempre più specifica formazione professionale di cui la medicina moderna necessita. Tutto ciò è comunque concepito nella consapevolezza che il disegno di legge n. 1142 sugli ordini qui in considerazione mira a istituire un migliore strumento di servizio a favore del cittadino, non a far nascere nuovi enti corporativi rinchiusi in deprecabili recinti autoreferenziali. Io penso che alla base di questa legge non vi sia tanto la la visione della nascita di nuovi enti, ma quella di andare ad individuare sempre più specifiche esigenze di salute che la medicina moderna richiede. Mi permetto di citare due esempi sulla nostra sanità che possono essere esplicativi di due ordini, quello degli infermieri e quello degli ostetrici. Ad esempio, per quanto concerne gli infermieri, riteniamo che sempre più la figura del laureato in scienze infermieristiche debba diventare responsabile del percorso clinico di un paziente.

si ha un abbattimento non solo dei costi ma anche della mortalità e della morbilità del paziente post-infartuato. Un altro esempio è quello del

una garanzia di specializzazione, di competenza, di modernità per la sanità italiana. [**Presidenza del

non vada d'accordo con la manovra che è stata appena varata da quest'Aula e che oggi dovrebbe approvare la Camera dei deputati, e, soprattutto, arrivi ad un punto in cui è invece opportuna una maggiore riflessione. Si dirà che sono decenni che si riflette: nel frattempo gli infermieri a suo tempo diplomati si sono laureati e chiedono giustamente di avere un riconoscimento ordinistico.

il mondo è cambiato.

alcune delle professioni che il passare degli anni ha visto profilarsi in modo diverso, più maturo, più radicato.

convinzione: è impensabile portare avanti questo provvedimento come se non ci trovassimo in una tempesta di crisi economica, che diventa crisi sociale e che ci impone di ripensare tutto il sistema ordinistico, e non non di aggiungere altri cinque ordini e venti albi professionali a ciò che già esiste. Mi chiedo come sia compatibile una scelta del genere con l'orientamento assunto dal dal Governo che, a corto di proposte dal punto di vista della crescita economica, ha detto, detto, scritto ed approvato con la manovra su cui ha posto la questione di fiducia che proprio l'accesso alle professioni deve diventare il primo tagliando per la crescita. Ma qui non stiamo facendo il tagliando per la crescita: stiamo piuttosto dando un altro taglio alla crescita. Mi permetta, signor Presidente, di fare alcune osservazioni per sollecitare maggioranza e opposizioni ad una riflessione che proprio il trascorrere del tempo dall'inizio dell'esame di questo provvedimento, con ciò che comporta, dovrebbe favorire. Mi permetto solo di portare una testimonianza: io mi sono trovato, come membro del precedente Governo,

vorrei fare un'osservazione di tipo generale, signor Presidente. Le esigenze sono reali. È evidente che, soprattutto nel campo delle professioni mediche e paramediche, ci troviamo di fronte ad abusivi, ciarlatani. Tra l'altro, l'uso della rete sta moltiplicando queste opportunità e questi rischi. Organizzazioni straniere anche a carattere illegale

Andiamo a vedere la sostanza del problema. Che ci siano delle esigenze reali è indiscutibile. Che esista la necessità di una regolamentazione leggera e non come questa, a mio avviso è altrettanto indiscutibile. Una regolamentazione leggera, e non quella contenuta nel provvedimento in esame, serve, signor Presidente, a dare le garanzie riguardanti la deontologia, la certificazione o la presa d'atto della formazione, riguardanti la tutela degli utenti e i controlli di qualità delle prestazioni che si fanno. Ma serve istituire 5 ordini e 20 albi per fare questo? Ma di che stiamo parlando?

Ma un fatto è disegnare il riordino delle grandi materie professionali in un contesto europeo e altro fatto è agganciare un ultimo vagone all'ormai deragliato treno della organizzazione degli ordini professionali negli ultimi sessant'anni.

professioni non vi sono limitazioni all'accesso, vuol dire garanzie per i giovani. Non è vero; non è detto che un ragazzo, se può ottenere un riconoscimento o un diploma o una certificazione

una dichiarazione di una tale chiarezza e nettezza da rendere impossibile al Senato approvare una simile misura.

il riscatto degli anni di studio per le professioni sanitarie, nel senso che si ammette al riscatto non il fatto di aver conseguito un diploma o una laurea, ma i periodi di studio per il conseguimento degli attestati. Ma vi è scappata la frizione? vi è scappata la frizione? e adesso volete dare la possibilità di riscattare degli anni di non si sa quali percorsi di formazione a fini previdenziali, anche

«come ampiamente già espresso nelle richiamate segnalazioni, si rileva che la costituzione di nuovi ordini professionali e dei relativi albi provoca una significativa restrizione della concorrenza, comportando limitazioni all'entrata di nuovi operatori, fatta eccezione per le ipotesi in cui, sussistendo un'asimmetria informativa tra consumatore e professionista, sia necessario, al fine di garantire maggiori benefici per i consumatori, consentire l'accesso a determinate attività

In assenza di tali presupposti, infatti, la previsione di forme di selezione all'entrata può comportare, sotto il profilo economico, un ingiustificato aumento dei costi dei servizi offerti, senza necessariamente garantire la qualità degli stessi».

di barriere all'accesso nel relativo mercato». A questo punto, signor Presidente, l'*Antitrust* si richiama a sue precedenti segnalazioni in cui, sotto il profilo della qualificazione professionale, si osservava che «le esigenze di tutela del consumatore possono essere integralmente soddisfatte con la previsione di un percorso formativo di livello universitario obbligatorio , come peraltro ribadito dalla Commissione europea da ultimo nella Relazione sulla concorrenza nei servizi professionali». dopo avere stigmatizzato il fatto che nella maggior parte degli Stati membri l'accesso alle professioni sia regolamentato con varie restrizioni, ha rilevato che una limitazione all'accesso al mercato si ripercuote negativamente sulla concorrenza e sulla qualità dei servizi, determinando un significativo aumento

Così stando le cose, signor Presidente, le chiedo di avanzare una riflessione all'Aula perché questo provvedimento venga reso radicalmente più leggero, ripensato e, comunque, non votato dal Senato della Repubblica, ma che anzi, a seguito di un approfondimento, possa tornare al nostro esame nelle settimane e nei mesi prossimi in una forma più seria e più credibile. Presidente, ho chiesto la parola, anche alla luce dell'intervento del senatore Rutelli, per riprendere la riflessione sviluppata ieri dal senatore Menardi nel tentativo di riproporre i temi che il senatore Rutelli ha ritenuto di sviluppare

e raccordarlo, renderlo conseguente, coerente, organico rispetto alle scelte che, da ultimo, in sede di manovra sono state fatte

della lotta all'abusivismo, del recupero di una qualità e di un'organicità in settori così fondamentali, tra l'altro con l'esigenza di raccordo

bisogna cercare di affidare alla Presidenza del Senato la scelta migliore, dal punto di vista procedurale, per salvare l'impostazione del lavoro che è già stato svolto e raccordarlo organicamente ad un disegno coerente che eviti una sorta di schizofrenia legislativa.

con la buona fede di chi ritiene che in ogni caso l'intervento riformatore sia necessario, anche se non nel modo e nelle forme previste, ovvero così dettagliatamente e con il rischio di una segmentazione delle professionalità, anziché in funzione di una riorganizzazione e di un recupero di organicità

né una dialettica Governo-opposizione. La verità è che esistono convergenze su talune impostazioni che attraversano la maggioranza come l'opposizione, così come esistono punti di criticità sulle medesime riflessioni che attraversano tanto la maggioranza

esame è un provvedimento di iniziativa parlamentare, segno di una risposta molto efficace, anche se articolata, della politica alle istanze di tanti professionisti che da oltre vent'anni attendono un atto di giustizia e di riconoscimento.

Il senatore Bosone ieri ricordava un aspetto molto importante: ci sono ragioni moderne su problemi antichi. E questo disegno d'iniziativa parlamentare in effetti pone un accento positivo su antiche diseguaglianze che si sono create nel mondo sanitario attraverso un ragionamento estremamente moderno ed attuale. Parlava anche della necessità di non lasciare al libero mercato la soluzione di questi problemi. Ed è tanto vero quello che ieri sosteneva in questa Aula il senatore Bosone che la Commissione europea non si è mai sognata di liberalizzare le professioni sanitarie. Infatti in tutta Europa sono tenute ampiamente fuori da questi ragionamenti, proprio perché la materia di cui stiamo trattando è estremamente delicata e complessa. Lo stesso ministro Fazio, nella penultima finanziaria, a domanda precisa da parte dell'opposizione, ha dichiarato: le professioni sanitarie sono fuori dal ragionamento di liberalizzazioni generali su cui il Governo si sta incamminando; proprio per essere attinenti alla storia italiana, ma soprattutto europea. Voglio anche ricordare,

passaggi parlamentari - che questi professionisti sono laureati; non hanno bisogno di esame di abilitazione, perché l'esame di laurea è automaticamente automaticamente abilitante e non c'è nessun blocco all'accesso. C'è asimmetria tra le conoscenze del sanitario e del pubblico. Ho ascoltato le critiche provenienti da alcuni colleghi, che non sono assolutamente fondate rispetto a queste professioni sanitarie, che non possono essere riconducibili ai ragionamenti che noi facciamo su altri Ordini quali gli avvocati o i notai. Sono due cose distinte ed hanno due percorsi abilitanti totalmente Non possiamo mischiare in questo *humus* generale aspetti diversi. E la parola di chiarezza di quest'Aula è fondamentale: una parola di chiarezza e di giustizia per questi professionisti. Tuttavia ieri mi è stata segnalata dalla senatrice Bassoli la necessità di riflettere su un argomento estremamente delicato, degno di grande attenzione. Ed anche gli uffici competenti mi hanno fatto rilevare questo c'è un punto della nostra legge che potrebbe creare conflitti di competenze sulla problematica delle sanzioni. In Commissione avevamo approvato, signor Presidente, un emendamento proveniente dal Gruppo dell'IdV, che prevedeva che che qualora l'ordine venisse a conoscenza di una situazione non corretta da parte del professionista, doveva far riferimento per le eventuali sanzioni agli organi competenti. Questa andata potrebbe creare

vero e delicato questo problema delle sanzioni, che ho detto alla senatrice Bassoli che vale la pena di riscrivere questa norma.

dopo avere io riscritto, come relatrice, un emendamento chiarificatore, il ritorno in Aula di questo provvedimento che, lo ribadisco, è stato votato in maniera unanime dalla Commissione sanità,

redigere un emendamento che risolva un problema posto dalla stessa relatrice. Ho ascoltato anche interventi più

mi limito a prendere atto di questa richiesta della relatrice. Se non vi sono obiezioni al riguardo, io accetterei la richiesta di sospensiva (perché non si tratta di un ritorno in Commissione, ma di una sospensiva del provvedimento); poi,

ha sollevato un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Procuratore della Repubblica

la motivazione della Camera -: «non spettava al primo esperire indagini nei confronti del deputato Silvio Berlusconi, Presidente del Consiglio dei ministri in carica, nonché compiere alcuni atti conseguenti, in tal modo precludendo alla Camera dei deputati l'esercizio delle proprie attribuzioni costituzionali in materia di cui all'articolo 96 della Costituzione; non spettava al secondo procedere in via ordinaria ed emettere il decreto di giudizio immediato nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, né affermare la natura non ministeriale del delitto contestato, omettendo di trasmettere gli atti al Collegio per i reati ministeriali». Con ordinanza 6 luglio 2011, n. 241, depositata in cancelleria il successivo 22 luglio, la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto e - ai sensi dell'articolo 37, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 ha disposto la notificazione del ricorso e dell'ordinanza stessa anche al Senato della Repubblica. Ricorso e ordinanza sono stati notificati al Senato in data 1° agosto 2011. Nella seduta del 13 settembre 2011, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, condividendo le argomentazioni contenute nel ricorso con cui la Camera dei deputati ha sollevato il predetto conflitto di attribuzione, ha espresso a maggioranza parere favorevole alla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica.

di intervenire in adesione al ricorso presentato dalla Camera dei deputati per sollevare conflitto di attribuzione nei confronti della procura della Repubblica presso il tribunale di Milano e del alla decisione di arrogarsi in via esclusiva il potere di decidere sulla natura del reato contestato al presidente del Consiglio, onorevole Silvio Berlusconi. L'adesione del Senato, ovviamente non obbligatoria ma certamente opportuna, si rende a nostro avviso necessaria per sostenere le ragioni di principio sollevate dalla Camera dei deputati in questa occasione, ma che certamente in futuro potrebbero riguardare Ministri appartenenti a questo ramo del Parlamento. Quindi, il Senato della Repubblica ha certamente interesse a intervenire per tutelare le prerogative del Parlamento. il ragionamento che svolge la Camera dei deputati è molto chiaro accettare l'interpretazione della Procura di Milano, e successivamente del GIP presso il tribunale di Milano, significherebbe accettare un'interpretazione assolutamente squilibrata e contraria al principio della leale collaborazione tra i poteri dello Stato. La legge costituzionale e la Costituzione stessa prevedono in modo esplicito che sulla natura del reato contestato ad un Ministro, tanto più al Presidente del Consiglio dei ministri,

una successiva valutazione più approfondita del tribunale dei Ministri e, infine, una valutazione non di ordine soltanto giuridico ma anche di opportunità politica del Parlamento. Se accedessimo all'interpretazione della Procura della Repubblica dovremmo accettare il paradosso che la Procura della Repubblica autonomamente

appartenenza del diritto-dovere di pronunciarsi in via definitiva sulla natura del reato. È un'interpretazione talmente dissociata e asimmetrica che non occorre un tecnico del diritto per capire che il conflitto di attribuzioni è non soltanto fondato, ma ha ragionevoli motivi di diritto per essere anche accolto. È anche un principio di buonsenso: nel nostro sistema costituzionale, formato di pesi e contrappesi, non c'è mai un organo che in via esclusiva può decidere per tutti inappellabilmente, ma c'è sempre un sistema di controlli, che invece in questo caso verrebbe assolutamente meno. Per queste ragioni, il Gruppo del PdL voterà a favore della Giunta, fermo rimanendo che qui non si tratta di stabilire, come ho sentito dire più volte, se nel merito

Qui si tratta semplicemente di stabilire se la Procura della Repubblica ha il potere esclusivo di decidere, da sola e senza alcun confronto con altro organo dello Stato, la natura del reato. Non siamo qui a sostenere che il reato sia di una natura piuttosto che di un'altra; noi sosteniamo che tale decisione competa in primo luogo al tribunale dei Ministri e in secondo luogo alla Camera di appartenenza, in un confronto tra organi e poteri dello Stato la natura stessa dei principi fondamentali su cui si basa la nostra Costituzione. Per tali ragioni, voteremo a favore

o in futuro, qualora attualmente non sia possibile (dalle informazioni che abbiamo assunto sembra che attualmente l'Ufficio per gli affari legali del Senato non disponga di una figura professionale abilitata all'esercizio

la legge costituzionale prevede in maniera esplicita che la decisione sulla ministerialità del reato compete alla Camera di appartenenza probabilmente è un auspicio di una legge che però non esiste. L'attuale legge non prevede questo.

il pubblico ministero, ossia l'organo dell'accusa, ha ritenuto la ministerialità del reato

la richiesta del pubblico ministero ritenendo che si trattasse di reato non ministeriale e quindi ha proceduto all'archiviazione sulla ministerialità trasmettendo gli atti per poi proseguire con il giudizio ordinario. In tale caso vi è proprio una previsione della legge costituzionale secondo cui, qualora vi sia l'archiviazione sulla ministerialità, bisogna darne comunicazione

nasceva una materia di conflitto, nel senso che, sollevato un problema di competenza, il giudice individuato, il tribunale dei Ministri, emetteva un provvedimento declinatorio della competenza; la legge costituzionale dice che in questi casi bisogna investire la Camera, e allora è ovvio che c'è una previsione nella legge costituzionale. Il caso al nostro esame rientra in tutt'altra ipotesi, l'ipotesi in cui l'organo dell'accusa non ha individuato la ministerialità del reato ma ne ha ritenuto l'ordinarietà, sicché il tribunale dei Ministri non è stato proprio investito della vicenda.

competente, ossia all'organo che esercita l'azione penale, stabilendo che, al posto di quella decisione se ne deve assumere un'altra, ossia quella della Camera di appartenenza, che diventerebbe organo dell'accusa. Questo è il paradosso giuridico: la Camera di appartenenza non promuove l'azione penale investendo un altro organo - perché quello è compito del procuratore della Repubblica - ma a quel punto cosa fa? Diventa organo d'accusa d'accusa investendo un giudice con la propria richiesta! Questo è veramente un paradosso giuridico. Io ho letto il ricorso che è stato fatto dalla Camera:

visto che siamo possibili litisconsorti, nel senso che la questione è comune ai due rami del Parlamento, avremmo diritto a costituirci in un giudizio che riguarda una materia che potrebbe interessare anche questo ramo del Parlamento. Senonché ci sono dei precedenti, e noi sappiamo, cari colleghi e onorevole Presidente, che il precedente è sempre stato la regola che ha ispirato i nostri comportamenti: si è sempre detto che esiste la prassi che vince sulla regola e la sostituisce, la interpreta oppure colma i vuoti regolamentari.

è rimasta totalmente indifferente. Non è mai successa una cosa del genere: dovremmo creare il precedente oggi. Finora avevamo avuto le leggi *ad personam*,

cerchiamo di essere lineari. Abbiamo dei precedenti parlamentari che non hanno visto la costituzione di un ramo o dell'altro del Parlamento in questa materia: continuiamo secondo le prassi! Perché dobbiamo cambiare il nostro comportamento, stratificato negli anni, per creare oggi un precedente? Ma che cosa diciamo agli italiani? Che spenderemo 20.000 o 30.000 euro soltanto perché dobbiamo

a questa costituzione in giudizio, che è offensiva per il diritto e i sacrifici che stiamo chiedendo agli italiani, sapendo che in questo modo andiamo a sprecare soldi che non sono nostri!

rappresenta, nel metodo e nel merito, un gravissimo esempio di strumentalizzazione a fini privati delle istituzioni e di profonda violazione delle norme che regolano i rapporti tra le funzioni e i poteri democratici nel nostro ordinamento. Anzitutto, la proposta della maggioranza nasce viziata in quanto si basa su di un assunto errato, e cioè che la procura di Milano, disattendendo la deliberazione

Secondo la maggioranza, infatti, avendo in quella sede la Camera statuito la natura ministeriale del reato (di concussione) ascritto al presidente Berlusconi, la procura di Milano avrebbe dovuto interrompere ogni ulteriore atto di indagine, spogliandosi del procedimento in favore del tribunale dei Ministri, il quale a sua volta avrebbe dovuto trasmettere gli atti alla Camera, per sentirsi formalmente negare (è questa la conseguenza inespressa ma coerentemente discendente dalla delibera) la possibilità di esercitare l'azione penale nei confronti del Presidente del Consiglio, ravvisando la sussistenza delle scriminanti della ragion di Stato o l'alta discrezionalità governativa Ebbene, tale assunto è radicalmente erroneo, in quanto omette di considerare che, in sede di autorizzazione *ex* articolo 68, secondo alla perquisizione domiciliare nei confronti del deputato Berlusconi (e non del presidente del Consiglio Berlusconi), la Camera non avrebbe certo dovuto (né potuto) pronunciarsi sulla diversa questione della natura ministeriale o meno del reato contestato: questo è un *ultra petita*. La Camera infatti può esercitare tale potere qualificatorio solo su iniziativa del tribunale dei Ministri, allorquando questo particolare giudice sottoponga la questione all'organo parlamentare, il quale non può, di propria iniziativa, pronunciarsi in ordine alla natura ministeriale del reato contestato. Se così non fosse, infatti, la Camera disporrebbe del potere di bloccare le indagini e paralizzare così l'esercizio della funzione giudiziaria, sol che un membro del Governo sia coinvolto in un procedimento penale. Si determinerebbe cioè una surrettizia reintroduzione dell'istituto dell'autorizzazione a procedere in relazione ai procedimenti a carico di Ministri o del Presidente del Consiglio. In secondo luogo, si ritiene che non sussista alcuna ipotesi di violazione delle prerogative della Camera. La proposta di maggioranza intende sollevare conflitto - nella forma della *vindicatio potestatis*

sancito che spetta esclusivamente all'autorità giudiziaria verificare i presupposti della propria competenza e cioè che è attribuzione esclusiva della magistratura

Nel merito, la proposta di elevare conflitto nei confronti dell'autorità giudiziaria (nella specie, la Procura di Milano) dissimula il tentativo di celare, sotto le vesti del conflitto interorganico, una mera strategia processuale della difesa del presidente Berlusconi, che finisce con il trasformare il Parlamento in una sorta di appendice del suo collegio difensivo, con una evidente strumentalizzazione delle istituzioni democratiche a fini meramente privati. del collegio difensivo del presidente Berlusconi. Infine, qualora la proposta della maggioranza venisse accolta, si darebbe corso ad un conflitto chiaramente inammissibile, in quanto sollevato in luogo di un mero conflitto di competenza; rimedio, questo, tipicamente endoprocessuale, che spetta alla difesa dell'imputato

innanzitutto occorre chiarire, al di là di quello che ho sentito, di cosa ci stiamo occupando. Ci stiamo occupando della costituzione del Senato in un giudizio per conflitto di attribuzione sollevato dalla Camera dinanzi alla Corte costituzionale, conflitto nei confronti della procura di Milano, che già è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale nel luglio di quest'anno. Ho sentito prima alcune affermazioni imprecise del senatore Li Gotti. Il caso Matteoli (è qui presente il ministro Matteoli e può confermarlo) è un caso recente nel quale il conflitto di attribuzione sollevato dalla Camera nei confronti del tribunale di Livorno ha visto poi la costituzione in giudizio in senso adesivo del Senato. Francamente (sono andato a rivedermi i resoconti delle sedute di Aula di quel periodo) non mi è parso di vedere senatori dell'opposizione che in quel caso si siano lamentati dell'intervento adesivo del Senato nel giudizio per conflitto di attribuzione sollevato dalla Camera nel caso Matteoli. Però qui, come al solito, quando viene fuori il nome di Berlusconi, ecco che allora anche le regole possono cambiare. Aggiungo poi che il ricorso sollevato dalla Camera nel caso Matteoli fu accolto dalla Corte costituzionale. La seconda motivazione che ci porta a votare a favore della proposta della Giunta è quella già indicata dal senatore Balboni. A chi spetta l'ultima parola in tema di ministerialità dei reati? A chi spetta stabilire se un reato sia o meno ministeriale? In questo caso la procura di Milano ha ritenuto di rubricare il reato di concussione telefonica - usiamo questa espressione tecnica - come reato comune e ha sottratto al tribunale dei Ministri e al Parlamento la conoscenza dei fatti relativi a queste ipotesi di reato, diminuendo oggettivamente le garanzie che la Costituzione, nell'articolo 96, prevede per i Ministri e anche - se l'opposizione consente - per il Primo Ministro Il problema sorge perché non esiste una definizione dei reati ministeriali nell'articolo 96, ma la dottrina più avveduta ha sempre sostenuto, senatore Li Gotti, che il principio di leale collaborazione porta a dire che, in caso di dubbio sulla natura ministeriale o meno di un reato commesso da un Ministro o da un Primo Ministro, debba esserci l'intervento immediato del tribunale dei Ministri, che non è un organo formato da politici compiacenti o da funzionari di partito: è un giudice formato da magistrati togati che fanno il loro dovere tanto quanto lo fanno i magistrati della procura di Milano e del tribunale di Milano. Dunque, il tribunale dei Ministri doveva essere immediatamente investito di questa ipotesi di reato da parte della procura di Milano, senza ritardo e senza compiere alcuna indagine. Così dice la legge costituzionale attuativa dell'articolo 96 e, soprattutto, il principio di leale collaborazione, che anche in questo caso salta quando si parla del Primo Ministro. Il tribunale dei Ministri avrebbe avuto 90 giorni di tempo - quindi non un tempo infinito, ma tre mesi per decidere sulla natura di quel reato: se avesse dovuto spogliarsi della competenza di quel reato inviando gli atti alla procura di Milano, con la cosiddetta procedura di archiviazione anomala, oppure se si trattava di un reato di natura ministeriale, che, quindi, doveva competere al giudizio del tribunale dei Ministri. si arriva a dire che il reato è stato compiuto sicuramente con abuso della qualità del Presidente del Consiglio, ma altrettanto sicuramente al di fuori di qualsiasi prerogativa del Presidente del Consiglio.

«sicuramente al di fuori di qualsiasi prerogativa del Presidente del Consiglio». Diventa davvero difficile seguire la procura di Milano in questo tentativo di evitare in tutti i modi l'intervento del Parlamento previsto su questo reato Ecco perché poi si alimentano gli eccessi di conflittualità tra politica e magistratura. C'è infatti qualcuno che del principio di leale collaborazione proprio non vuole sentire parlare. LNP)*. Pertanto, i dubbi in ordine alla natura ministeriale di questo reato, e credo che siano i dubbi che la stessa lettura del decreto del GIP evidenzia chiaramente, dovevano portare tutto al tribunale dei Ministri.

per tutti gli altri casi che si potranno porre in futuro e che magari un giorno interesseranno anche ministri dell'attuale opposizione. Quindi, proprio per questi motivi il nostro voto sarà favorevole all'approvazione

A me non sembra. A me sembra che questo interesse nasca dal fatto che la tutela data ad un membro del Governo per un reato ministeriale poi porta questa Camera, il Parlamento, ad essere giudice che può eliminare il reato, anche se il reato è evidente e non è ministeriale. E questo è stato già sperimentato, in maniera del tutto inappropriata. Vorrei dire ai colleghi che abbiamo una responsabilità importante questa responsabilità è quella di non abusare delle tutele costituzionali, perché quando questo abuso c'è, poi il Paese ce la fa pagare e non riconosce più la credibilità e l'importanza del Parlamento e toglie le tutele alla funzione parlamentare. Stiamo attenti a quello che facciamo anche oggi. I Capigruppo di maggioranza della Camera, per sostenere la levata del conflitto di attribuzioni, hanno detto che il Presidente del Consiglio ha chiesto informazioni ad "un dipendente della Questura" (è scritto così nella lettera al presidente Fini). Invece, quel che abbiamo saputo, anche nelle carte consegnateci, è che ci furono pressioni perché una signorina minorenne - dico il nome perché non si è ancora pronunciato in quest'Aula, forse per un pizzico di pudore ipocrita - Karima El Mahroug, nota "Ruby Rubacuori", in stato di fermo presso la questura di Milano, fosse rilasciata ed affidata ad una persona che non aveva qualità per essere affidataria di questa minorenne, la signora Nicole Minetti. Bene, il procuratore è un semplice passacarte in questi casi? È un passacarte al tribunale dei Ministri, come abbiamo sentito essere sostenuto? No. solo se il reato è ministeriale. E la condotta posta in essere dal Presidente del Consiglio - perché è di questo che dobbiamo occuparci oggi ha una qualche attinenza con il suo compito di "dirigere la politica generale del Governo", come è detto nella nostra Costituzione? La risposta è no. Allora, a meno di non dover aderire alla tesi difensiva per la quale il Presidente del Consiglio si batteva per evitare un grave incidente diplomatico in quanto la signorina El Mahroug era - così gli constava la nipote dell'allora presidente egiziano Mubarak, noi dovremmo dire no alla sollevazione del conflitto di attribuzione. Perché il Senato, elevando il conflitto, esplicitamente finisce per aderire a questa che chiamerei "mozione del ridicolo". Può il Senato ridursi al personaggio credulone di questa triste e fangosa commedia? Penso di no. Ciascuno di noi e ciascuno di voi risponda a questa domanda e ricordi che ha, per la sua parte, la responsabilità di difendere la dignità e la collocazione costituzionale del Parlamento. C'è, infine, una raccomandazione della Giunta, questa sì, votata all'unanimità perché il Senato, se decide di costituirsi - e noi riteniamo che non si debba costituire - lo faccia direttamente - come ha diritto di fare - senza oneri a carico del suo bilancio. Se non ci si salva l'anima, almeno non si intacchi la cassa.

se cioè non ci rendessimo conto che stiamo discutendo e votando su una questione di merito, che riguarda quello che è stato definito anche in questa Aula come una ipotesi di reato di concussione telefonica, e capire se questo reato di concussione telefonica sia ordinario o ministeriale, ci arrampicheremmo sugli specchi. è oggettivamente difficile e complicato far passare all'opinione pubblica mondiale e italiana l'idea che la telefonata fatta dal *Premier* per far rilasciare una signorina con la quale si accompagnava in altre faccende sia una questione ministeriale. Oggettivamente è un qualcosa che va oltre il buon senso. Ma Ma se anche volessimo eliminare la discussione di merito nel suo complesso e fare una valutazione più oggettiva, è complicato spiegare

la scheda istruttoria che accompagna qualsiasi atto in questo Senato. Non sappiamo che cosa ha costruito l'altro ramo del Parlamento. Non si capisce perché il Senato si debba costituire, anzi si capisce: c'è un solo ed unico obiettivo, quello di poter dire ai decisori che, oltre alla Camera, anche il Senato - quindi, in qualche modo, tutta la politica - solleva il conflitto di attribuzione. Non è così. Non è tutta la politica, anzi ci sono una buona parte della politica, almeno quella che riguarda il mio Gruppo, e la stragrande maggioranza dell'opinione pubblica che non capiscono perché si solleva questo conflitto di attribuzione. Anche per questo - soprattutto per questo - non possiamo essere d'accordo sulla deliberazione che ci viene proposta. Signor Presidente, se il Senato votasse favorevolmente la partecipazione al giudizio per il conflitto di attribuzione credo commetterebbe un abuso,

il Senato dovrebbe associarsi a questo conflitto di attribuzione. Ho sentito poi l'intervento del senatore Mazzatorta, e mi sembra che tutti gli interventi finora svolti girino intorno ad una questione inequivoca dal momento in cui, nel 1989, l'articolo 96 della Costituzione è stato riformato. L'articolo 96 della Costituzione dice che i Ministri e il Presidente del Consiglio dei ministri sono sottoposti alla giurisdizione ordinaria, e la legge costituzionale, che attua la previsione costituzionale, dice che la Camera di appartenenza - esclusivamente la Camera di appartenenza

due scriminanti, che sono di natura squisitamente politica: l'essere cioè il fatto reato commesso nell'esercizio di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante o per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione. Il fatto è reato ma viene scriminato da queste due ragioni, ragioni, che sono due vere e proprie scriminanti di natura e di rilievo politico-costituzionale. Tutto il resto del procedimento, dall'individuazione del fatto ascritto come reato ministeriale in poi, è materia che appartiene alla giurisdizione ordinaria e viene regolata anche nella relazione tra il cosiddetto impropriamente tribunale dei Ministri, composto da giudici ordinari, e il procuratore della Repubblica, ed eventualmente il GIP, dalle regole ordinarie del codice di procedura penale in materia di competenza. Ripeto, in materia di competenza. La La inscrivibilità di un fatto nell'ambito dei reati ministeriali o meno appartiene integralmente al procuratore della Repubblica che riceve l'atto, e lo fa sulla base di una giurisprudenza consolidatissima, oltre che della lettera della Costituzione. Esiste una bella differenza, senatore Mazzatorta, non fumosa - biblioteche sono dedicate al tema - fra un fatto commesso nella qualità e un fatto commesso nell'esercizio delle funzioni. È sulla base di questo criterio di orientamento, della molteplicità delle fonti giurisprudenziali e normative che disciplinano detta differenza, che la magistratura Se il tribunale dei Ministri ritiene che invece sia competenza propria, promuove un conflitto di competenza. Il conflitto di attribuzione è del tutto destituito di fondamento.

una "marchetta" nei confronti del Presidente del Consiglio: un ulteriore espediente per allontanare il tempo in cui dovrà rispondere al suo giudice PD).*Ritardo che gli è congeniale, ma poiché è tanto affezionato all'idea della libertà personale (così tanto e così spesso la invoca) dovrebbe da teste andare a rendere la propria testimonianza, perché ogni ora di remora è un'ora in più di restrizione per la libertà personale di due persone che in questo momento sono in carcerazione preventiva in quanto imputati di un reato di cui il Presidente del Consiglio è parte offesa. Allora finiamolo, smontiamolo questo castello di imprecisioni, di fumisterie e di forzature, perché in tutto questo chi ci perde è l'istituzione che in questo momento noi, per caso, rappresentiamo: è la sua dignità, la sua autorevolezza, il suo rango, il suo rango nell'ordinamento. Non è quindi per ragioni di avversione politica: è per ragioni che tentano di restaurare la la dignità del lavoro che facciamo e il prestigio di questo ramo del Parlamento che noi voteremo assolutamente no al fatto che il Senato si associ al conflitto di attribuzione. Presidente, onorevoli colleghi, il mio intervento sarà assolutamente breve, dopo l'ottimo e puntuale intervento svolto dal collega Li Gotti, che ha affrontato, con la maestria che gli è propria, il profilo tecnico-giuridico della materia. Voglio motivare il no del Gruppo dell'Italia dei Valori sotto un profilo politico e morale. morale. Sempre il collega Li Gotti dichiarava ieri che il senso del ridicolo, purtroppo, non è ancora colto per intero dalla maggioranza dei colleghi, in particolar modo dalla maggioranza che siede qui in Senato.

potente presidente dell'Egitto, poi evidentemente colpito dal malocchio per essere stato trascinato in questa vicenda, significa coprire le istituzioni e il Senato del senso del ridicolo. L'Italia dei Valori vi chiede di evitare questa ennesima buffonata. *(Applausi Sappiamo bene quali sono le vicende che collegano la signorina Rubacuori a Tarantini, a Lavitola, Lavitola, e potremmo continuare la costellazione di riferimento del Presidente del Consiglio, che non hanno niente a che vedere con il conflitto di attribuzioni. Vi prego allora di evitare questo sciagurato errore che alla fine ricadrà, come sta ricadendo, per intero anche sulla parte buona che nel centrodestra ancora c'è. Fermatevi sulla soglia dell'ennesimo burrone per evitare di precipitarvi ancora una volta.

da parte dell'autorità giudiziaria, la qualificazione in ordine alla ministerialità o meno del reato e in che misura e in quale fase questa qualificazione viene condotta, e se c'è una garanzia da parte del Parlamento in ordine ad un successivo apprezzamento e ad una successiva valutazione. Se soffermiamo l'attenzione su questi aspetti e, in particolar modo, oltre che sull'articolo 96 della Costituzione, sulla legge costituzionale n. 1 del 1989, che ha delineato il relativo procedimento, ci rendiamo conto da subito, se la norma viene letta con occhio scevro da pregiudizio e in maniera assolutamente serena, che alla procura della Repubblica, una volta pervenuta la *notitia criminis*, non compete alcuna funzione né è riconosciuta alcuna attribuzione in ordine alla qualificazione del reato, perché la norma testualmente impone l'immediata sospensione di ogni attività e la remissione degli atti ad un altro organo giurisdizionale, ovvero il tribunale dei Ministri. deve - entro un termine correttamente ricordato dal senatore Mazzatorta - pronunciarsi nei 90 giorni dalla remissione della questione.

perché in quell'occasione la deliberazione assunta da questa Assemblea (luglio 2009) ha focalizzato un punto centrale rispetto all'esame della sequenza procedimentale, vale a dire rispetto addirittura alla funzione del tribunale dei Ministri

che compito del tribunale dei Ministri è condurre un istruttoria, una qualificazione e poi, comunque, le risultanze rassegnate devono vedere in una fase successiva un necessario coinvolgimento del Parlamento.

Gotti. Questa sentenza afferma un principio fondamentale rispetto alla vicenda che stiamo esaminando. In essa si afferma che all'organo parlamentare non può essere sottratta una propria autonoma valutazione sulla natura ministeriale o non ministeriale dei reati oggetto di indagine giudiziaria, né tanto meno, ove non condivida la conclusione negativa espressa dall'autorità giudiziaria, la possibilità di sollevare un conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale, assumendo di essere stata menomata per effetto della decisione giudiziaria della potestà riconosciutale dall'articolo 96 della Costituzione. Quindi, la posizione del Parlamento non è né potrebbe essere una posizione neutra, proprio perché stiamo parlando della tutela di una prerogativa del Parlamento. Questo principio peraltro é pacificamente condiviso: mi permetto di ricordare che proprio nel caso che stiamo trattando è la stessa procura della Repubblica di Milano che, nella memoria consegnata nel giudizio relativo al conflitto di attribuzione, ha espressamente richiamato questo principio, fissato nella sentenza della Corte costituzionale, sostenendo che se il Parlamento si doleva di questa iniziativa intrapresa dall'autorità giudiziaria e la riteneva non conforme al dettato costituzionale e alla legge costituzionale n. 1 del 1989, avrebbe dovuto attivare il rimedio del conflitto di attribuzione. Ed è esattamente ciò di cui stiamo discutendo. Mi permetto anche di osservare, in relazione all'intervento della presidente Finocchiaro, che la decisione di spiegare l'atto di intervento nel giudizio sul conflitto di attribuzione da parte del Senato è qualcosa che deriva dalla legge che disciplina il giudizio dinanzi alla Corte costituzionale, la quale impone la notifica ad entrambi i rami del Parlamento che il nostro sistema costituzionale - come è ben noto a tutti - è fondato sul principio del bicameralismo perfetto. Quindi, in sostanza, la tutela delle prerogative del parlamentare interessa il Parlamento nella sua pienezza e totalità e non solo il ramo al quale appartiene. È questa la *ratio* per la quale è prevista la notifica, ed il suo effetto, cioè la conoscenza legale dell'esistenza di questo giudizio, è la possibilità offerta al soggetto destinatario della notifica, al pari di quanto avviene in qualsiasi altro procedimento giurisdizionale, di promuovere un proprio intervento, che in questo caso è di natura adesiva rispetto al conflitto sollevato dalla Camera dei deputati. Quindi, non è una stravaganza, una iniziativa o una forzatura del sistema: siamo nella dinamica fisiologica del rapporto processuale. D'altra parte, che questo sia vero è confermato anche dai tanti precedenti che sono stati ricordati in ordine alla costituzione di entrambi i rami del Parlamento. E se mi è consentito, proprio rispetto alla posizione dei Ministri, che il Senato abbia, pur nel rispetto del principio del bicameralismo perfetto e quindi della parità tra i due rami del Parlamento, una posizione per così dire rafforzata deriva dalla previsione della legge costituzionale che attribuisce proprio al Senato della Repubblica, nel caso in cui il Ministro non sia parlamentare, la competenza a pronunciarsi su questa materia. Quindi, noi siamo un organo Vorrei aggiungere, una considerazione anche rispetto all'affermazione resa nell'intervento della presidente Finocchiaro a proposito della competenza

davvero *in claris non fit interpretatio* - cessa ogni azione investigativa di indagine immediatamente e, subito dopo, c'è da parte del tribunale dei Ministri, altra autorità giudiziaria, la competenza a svolgere un apprezzamento specifico su questo profilo. noi correttamente manteniamo il dibattito in questo alveo, ci rendiamo conto che il Senato ha un suo interesse, perché stiamo difendendo una prerogativa del Parlamento.

costituzionale, che ha rimarcato come ci sia una necessaria autonomia del Parlamento nella valutazione della ministerialità del reato: l'effetto di quanto accaduto nella vicenda che stiamo esaminando è è che, proprio per l'iniziativa indebita, quella sì, illegittima della procura della Repubblica, al Parlamento di fatto viene sottratta la possibilità di condurre in maniera autonoma questo apprezzamento e questa valutazione. Quindi, difendiamo una prerogativa del Parlamento e non entriamo nel merito della vicenda, perché noi non dobbiamo giudicare in ordine alla telefonata, alla valenza probatoria di quella telefonata, a tutte le ragioni che sono connesse a questi aspetti, ma dobbiamo difendere un sacrosanto principio che è appunto quello di garantire la la corretta applicazione di una norma costituzionale, di una legge costituzionale, che sono a presidio di un valore di importanza assoluta in un sistema democratico e parlamentare quale è appunto il nostro. Credo che il Senato debba opportunamente intervenire in questo giudizio, spiegando l'intervento adesivo. Mi permetto di osservare che, proprio per la complessità della questione e per l'alto valore giuridico della vicenda, è necessario che questa rappresentanza del Senato sia affidata, secondo l'ordinamento vigente e le disposizioni che disciplinano

ricordando a me stesso innanzitutto che quello dinanzi alla Corte costituzionale è un giudizio che anche dal punto di vista formale richiede una competenza e un'attenzione del tutto particolari. Pertanto, difendiamo un valore del Parlamento, e difendiamolo bene, affidandolo a persona professionista che sia decisamente all'altezza del compito.

«raccomanda, altresì, che la costituzione in giudizio, al fine di non gravare, con le relative spese, sul bilancio del Senato, avvenga nelle forme dell'intervento diretto e della comparsa personale prevista dagli articoli 20 e 37 della legge n. 87 del 1953».

allo stato, non è dotato di professionisti abilitati presso le magistrature superiori. Io raccolgo, comunque, l'invito del senatore Balboni a porre in Consiglio di Presidenza la soluzione eventuale di questo tema, attraverso un eventuale rimpinguamento di quelli che sono i ruoli dell'Ufficio affari legali del Senato. È un tema che, naturalmente, discuteremo in Consiglio di Presidenza nella logica della riduzione dei costi complessivi del Parlamento.

una risposta affermativa, nel senso di dotare il Senato di una possibile competenza che intervenga anche in giudizi di questo tipo. Io ritengo, però, per evitare qualsiasi equivoco

di fronte alla Corte, in questo caso deve essere rappresentato da un professionista, così come prevede la legge e così come prevedono la complessità e la serietà della materia che stiamo trattando.

Quando la legge di organizzazione della Corte costituzionale dice che gli organi costituzionali possono stare in giudizio davanti alla Corte direttamente e personalmente, secondo me non prescrive che il Senato o la Camera dei deputati si dotino di una struttura abilitata al patrocinio, bensì configura il privilegio, dato all'organo costituzionale, di presentarsi anche con una memoria dell'organo politico

Signora Presidente, è scomparso Walter Bonatti. La sua morte non può non colpire l'intera comunità nazionale, ancora memore del suo sacrificio sul K2 per consentire a Compagnoni e Lacedelli di piantare su quella cima la la bandiera italiana. Seguirono polemiche roventi dalle quali Bonatti uscì con il profilo leale, cristallino e battagliero che ha caratterizzato la sua avventura umana: perché di avventura si tratta, se solo si pensa alle eroiche ascese invernali e ai suoi indimenticabili *reportage* sul settimanale "Epoca". Alpinista, esploratore, scrittore, uomo soprattutto curioso e di fascino contagioso. Amava Lecco, la mia città, e le guglie della Grigna, che frequentava con la stessa disinvoltura con la quale noi facciamo due passi in centro. Viveva nella vicina Valtellina, ma era sempre in giro per il mondo a scrutare e raccontare. Mancherà a tutti questo personaggio, il suo punto di vista, il suo occhio sul mondo, ma soprattutto avremo nostalgia di un gigante della montagna onesto e innamorato della natura. Alla famiglia, in particolare alla moglie Rossana Podestà, la vicinanza di tutto il Gruppo Lega Nord del Senato e di chi come me ha avuto l'onore di conoscerlo.

qualche mese è in corso un'agitazione per l'annuncio di una ristrutturazione industriale e di una vendita del sito; inoltre, da settimane

della Valle dell'Ufita, in provincia di Avellino, è l'unico stabilimento in Italia ad avere il *know-how* specifico per la produzione dei pullman. dunque, di una decisione che ha gettato nello sconforto - come si può immaginare - i lavoratori ed i cittadini di quel territorio. Pertanto, chiediamo al Governo

che vorrei ricordare con una sua frase. Diceva Zizola: «Osservare, analizzare e raccontare queste vicende, spesso avvolte nel segreto, non era facile. Per questo il compito dell'informazione divenne, a partire dal Concilio Vaticano II, un capitolo nevralgico non privo di contrasti e di agguati per mettere alla prova la conclamata riconciliazione della Chiesa con le libertà moderne». Penso sia importante ricordarlo.

nei giorni scorsi organi di informazione hanno ripreso il comunicato stampa di un sindacato di Polizia denominato COISP, il quale prendendo spunto dai famosi prezzi del ristorante del Senato - di cui peraltro in quel momento era già stato deciso il drastico aumento

via. Innanzi tutto, questa vicenda è l'indice di una campagna di odio sistematico che viene diffusa su molti organi di informazione,

attenzioni particolarmente negative, ai limiti dell'aggressione, mi pare persino di rilevare un certo compiacimento, come per dire «stiamo riuscendo nella campagna». Io non credo che si debba aspettare il momento in cui ci saranno delle aggressioni personali violente vere e proprie per prendere delle posizioni. Non credo che possiamo tollerare oltre di ascoltare passivamente queste cose, specialmente quando sono infarcite sistematicamente

Io credo che sia giunto il momento di intraprendere azioni legali e anche di altro tipo per avere una tutela. In particolare - e torno al primo episodio di cui ho parlato - è inquietante che delle persone che hanno il delicato e difficile incarico di tutelare l'ordine pubblico, per il quale loro stessi, anzi loro per primi, a trovarsi di fronte a manifestazioni violente e ad esserne le prime vittime, cosa che giustamente quel sindacato sottolinea con forza chiedendo ogni tutela possibile (ed è nostro assoluto dovere dare loro solidarietà in modo concreto e prevedere ogni tipo di tutela), persone, dicevo, che hanno un incarico così delicato, parlino di sparare contro contro il Senato. Trovo che sia veramente inaccettabile, e guarda caso i giornali di oggi, quando l'hanno riportato, hanno totalmente ignorato le reazioni che da parte di alcuni - pochi - parlamentari ci sono state a seguito

volantino per quello che è, e non credo che tutti i poliziotti abbiano lo stesso pensiero.

ho letto su «Il Sole 24 Ore» che l'AIFA sta dando l'autorizzazione alla commercializzazione del farmaco detto pillola farmaco si hanno due diverse idee: per chi, come me, crede che la vita inizi all'inizio del concepimento è una pillola abortiva; per molti è una pillola anticoncezionale.

che i giornalisti - come tutti quelli che abbiamo affrontato oggi - appartengono ad un ordine professionale. Si dimostra quindi l'inutilità dell'ordine, anzi, se possibile, l'ulteriore garanzia dell'impunibilità degli stessi, ferma restando la libertà di espressione del migliore o del peggiore dei sindacati della Polizia. Posto che, chiaramente, è nella disponibilità di chiunque adire le vie legali nei confronti di qualcuno, tengo a sottolineare che dovremmo avere a che fare con l'ordine dei giornalisti per ricordare come questi signori non solo, come ha detto la Presidente, facciano di tutta l'erba un fascio, ma sicuramente

a seguito di due o tre anni di campagna quotidiana sistematica contro le istituzioni, occorrerebbe vedere finalmente utilizzati quei soldi per una operazione di verità: non dico di difesa, perché sappiamo che non dobbiamo difendere noi stessi dal doveroso rendere quanto più possibile fruibili i dati relativamente a ciò che quotidianamente viene utilizzato per attaccarci. Queste erano le due uniche questioni che credo debbano essere ricordate quando si parla del

qualunquista al qualunquismo che attacca Camera e Senato quotidianamente. Signora Presidente, vorrei aggiungere alle parole di preoccupazione espresse dal senatore Malan alcune brevissime considerazioni.

sia in realtà un aspirante politico, perché più volte candidato ad elezioni in svariate situazioni. Penso anche che uno dei punti che andrebbe messo in evidenza è quanta poca trasparenza esista all'interno di queste organizzazioni sindacali dal punto di vista della rendicontazione, dei loro bilanci e dei loro reali iscritti. Ma la cosa più grave - ed è il motivo del mio intervento e della mia accorata richiesta a lei, signora Presidente Presidente - è che questa espressione giunga da un appartenente alle forze di Polizia e dell'ordine, cioè una persona che dovrebbe essere garante della legalità e del rispetto anzitutto delle istituzioni, in particolar modo quelle democraticamente elette dal popolo italiano. Chiedo quindi a lei, signora Presidente, di farsi promotrice di una richiesta al ministro dell'interno Maroni perché di questo possa venire a rispondere in Parlamento, alla luce delle per quanto rare stigmatizzazioni già pervenute dai rappresentanti del Parlamento: è di ieri quella del Partito Democratico, è di oggi, in Aula, quella del senatore Malan per il PdL. Vorrei aggiungere aggiungere la richiesta al Ministro - che anticipo sarà oggetto di una mia interrogazione parlamentare - di riferire su quanto si apprende oggi, leggendo la stampa quotidiana, a proposito di un'importante e quanto mai inquietante denuncia da parte di un agente dei NOCS rispetto ad un clima e alla pratica, che pensavamo aver dimenticato e sepolto nella nostra memoria, del nonnismo all'interno di questo corpo speciale. Ricordo che dovrebbe essere una delle punte di eccellenza della nostra sicurezza, della lotta al terrorismo ed alla grande criminalità, ed invece si macchia, ovviamente fino a quando non sarà fatta piena luce su questi fatti, di abusi, quasi sempre a sfondo sessuale, di vere e proprie molestie, compiute davanti a numerosi testimoni, che evidentemente, a causa dell'obbligo omertoso, coprono con il loro silenzio pratiche di questo genere. Auspico che il PM Elisabetta Ceniccola, che sta svolgendo queste indagini, possa farlo nella massima trasparenza possibile, che il ministro Maroni sia garante di questo e che lo stesso possa rispondere in quest'Aula di come può accadere che un poliziotto ed un rappresentante

sia attraversato da questi fenomeni e sia animato da personaggi del genere. Mi auguro e auspico che l'inchiesta della procura di Roma possa mettere in evidenza tutta la sua verità e possa tranquillizzare i cittadini italiani e il Parlamento italiano rispetto ad un clima pericolosissimo che si sta addensando attorno alle forze di Polizia nella relazione e nel rapporto tra esse e il Parlamento, e il Parlamento, tra esse e lo Stato italiano e i cittadini italiani.

viste le preoccupazioni che sono state sollevate da parte di vari colleghi, veramente sento il dovere di esprimere la mia grande preoccupazione preoccupazione per l'immagine di istituzioni che noi stiamo rappresentando, e con questo anche per la stessa democrazia, che si sta mettendo in gioco in questi giorni. Signora Presidente, la prego pressantemente di coinvolgere la Presidenza di quest'Aula, insieme con la Presidenza della Camera, per affrontare il problema dell'immagine pubblica della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e dei membri di queste due

forze sommerse cercavano di mettere in pericolo la democrazia per tutti altri interessi. Signora Presidente, leggiamo sulla stampa e su Internet articoli indecenti pieni di falsità. È stato citato quello del sindacato dei poliziotti, ma questo è solo uno dei tanti Mi metto in prima fila e ci mettiamo tutti in prima fila quando si tratta di ridurre i costi della politica, ma su tale aspetto, per esempio, non è stato pubblicato quello che è stato fatto seriamente dal Parlamento stesso,

intervengo per avanzare una proposta, condividendo le analisi svolte da molti colleghi. Mi permetto di raccontare all'Aula un piccolo episodio personale. Per vicende personali e familiari, a metà agosto

reparto stava morendo e parlavano di noi, definendoci «delinquenti» e specificando i costi di ogni piatto.

ma verso questi organi costituzionali della rappresentanza. E quando gente molto perbene (titolare di piccole imprese, professionisti, lavoratori) si arrovella su questi particolari,

hanno ragione i colleghi che hanno detto che se un singolo parlamentare invia una lettera ancora lo sbertucciano, ma io chiedo una cosa molto semplice:

un quarto di pagina del «Corriere della Sera» o de «La Stampa» e di volta in volta svolga un lavoro di informazione e di monitoraggio sulle piccole o grandi cose che stiamo facendo.

Presidente, intervengo a seguito dell'intervento della senatrice Spadoni Urbani che ha sollecitato la possibile discussione di una mozione sulla

al di là del fatto che ciascuno può credere che la pillola sia una cosa o un'altra, esistono delle evidenze scientifiche che, invece, sono cosa diversa dai pareri e dalle opinioni personali. La pillola dei cinque giorni dopo è un contraccettivo di emergenza

Il lavoro che avrebbe dovuto fare AIFA, la nostra Agenzia del farmaco italiano, era semplicemente quello di recepire la decisione europea e di commercializzare il prodotto in Italia. L'AIFA si sarebbe dovuta limitare, con la procedura di prassi di 90 giorni, a stabilire il prezzo, la rimborsabilità ed eventualmente la prescrizione con ricetta medica. Peccato che l'AIFA faccia anche un altro vero lavoro: quello di assecondare le opinioni, che sono cosa diversa dalle evidenze scientifiche.

caso, il Consiglio superiore della sanità ha dovuto rispondere alle evidenze scientifiche, però ha aggiunto che avrebbe potuto anche diventare un abortivo nel caso in cui la donna fosse incinta.

che prima di assumere un contraccettivo di emergenza, la cui azione al massimo può essere esaustiva nel tempo di cinque giorni da un rapporto sessuale

sarebbe l'impianto meraviglioso creato, appunto, per assecondare le opinioni e le idee di chi crede che questo sia un farmaco abortivo e non un contraccettivo. tolto tutto questo, è dal mese di febbraio 2010 che l'Agenzia italiana del farmaco deve espletare una richiesta di autorizzazione in commercio di un farmaco riconosciuto a livello nazionale e internazionale come contraccettivo d'emergenza. Abbiamo presentato l'interrogazione in questione e mi auguro che ci sia data risposta, ma soprattutto che in Italia si smetta davvero di confondere le opinioni personali con quelle che sono le evidenze scientifiche.

a proposito dell'antipolitica e dei poteri forti, delle agenzie di *rating* e dei banchieri centrali che definisco

fonte di quella tabella nella quale ci fanno passare per ladri. Non mi sento di appartenere alle caste, ma ritengo che bisogna reagire. reagire. Se la politica è debole e in una fase come questa è debole, sono altri che surrogano la funzione nobile della politica di difendere gli interessi generali di tutti,

Moody's, Standard & Poor's e Fitch Ratings, continuano ad emettere rapporti ad orologeria sui debiti degli Stati, pur senza che ci siano le richieste, facendo quindi deprimere il valore delle azioni, delle obbligazioni e dei titoli di Stato. Ebbene, c'è una inchiesta della procura di Trani, e al riguardo ho presentato molte interrogazioni, che ha rinviato a giudizio l'amministratore delegato di Standard & Poor's, quella stessa agenzia che ha declassato il debito americano non accorgendosi di un errore di 2.000 miliardi di dollari. ha fatto un errore di 2.000 miliardi di dollari. che questa cricca del *rating* in Italia non è registrata all'ESMA, ossia l'ente europeo

o di Draghi ma è del popolo italiano, sempre per ridurre il debito pubblico. La questione è che la politica, se non vuole essere ostaggio di questi signori, deve reagire

emettere rapporti né sull'Italia, né sulle aziende italiane. Non sarebbe sbagliato se istituzioni come il Senato potessero far sentire la propria voce, se le istituzioni

seduta per ricordare come prima di grandi tragedie del secolo scorso grandi filosofi, come Oswald Spengler, avevano criticato la democrazia e la sua corruzione ed attaccato la Repubblica di Weimar.

Ma voglio aggiungere un altro elemento fondamentale. Forse noi politici dovremmo fare un po' di autocritica e pensare quello che pensa, in realtà, la stragrande maggioranza dei parlamentari (perché dobbiamo cominciare a dire anche questo). La stragrande maggioranza dei parlamentari svolge il suo mandato di rappresentanza con spirito di servizio nei riguardi del Paese e degli interessi superiori del Paese; però, ogni tanto vengono commessi o grandi abusi, come nel caso di colleghi che con la sirena si fanno scortare superando le code, o guidando nella corsia di emergenza in autostrada. Sono queste cose le cose

nazionale. Abbiamo di fronte uno scenario assolutamente plausibile e possibile di riforme condivise, perché i cittadini saranno in grado di condividerle.

dalla mafia e dal terrorismo. Non deve stupire se un piccolo o grande dirigente di un sindacato si esplicita alla sua piattaforma sindacale anche attraverso forme violente. Non ci dobbiamo meravigliare, perché questo fa parte della democrazia, e se queste critiche sono state espresse sopra le righe esistono gli anticorpi per correggerle. Credo, quindi, che l'intera vicenda debba essere riportata all'interno di un alveo che deve necessariamente portare i parlamentari e il Parlamento ad affrontare questi temi con spirito non corporativo, ma aperto, perché la democrazia è soprattutto lotta di idee e, anche critica delle sue disfunzioni. *(Applausi